L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Onorevoli colleghi, la Camera dei deputati ha approvato con modificazioni e trasmesso il disegno legge di conversione del decreto-legge in materia di autotrasporto,

alla Commissione di merito di riferire all'Assemblea nella giornata di domani, come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo. Gli emendamenti dovranno essere presentati entro le ore 11 di domani.

e del rendimento delle strutture pubbliche e dei loro dipendenti. Delega al Governo in materia di valutazione del rendimento delle pubbliche amministrazioni e del loro personale ed in materia di responsabilità dei dipendenti pubblici***

che riprendono dei temi accennati genericamente nelle precedenti normative. Noi vogliamo responsabilizzare la dirigenza

si muove nella stessa direzione. In particolare, noi riteniamo che la valutazione obiettiva dei risultati e il premio al merito, che è questione generale, valgano anzitutto

a verifica, alla luce di criteri obiettivi che si ispirino al merito e alla capacità di assumere stessi. Sottolineo l'importanza di questi due emendamenti. Grazie per l'attenzione.

e inoltre si sopprimerebbe la disciplina del conferimento di incarichi a soggetti estranei. Quanto all'emendamento 5.301, che è stato illustrato poco fa dal senatore Izzo,

vorrei chiedere al relatore in quale parte del testo che stiamo esaminando è ricompreso il contenuto dell'emendamento 5.19,

Presidente, nei cinque minuti di sospensione ho potuto esaminare e confrontare il testo dell'emendamento 5.19 con l'articolo 6, comma 2, mi sono fatto la convinzione che il contenuto di questo emendamento ben implementa e completa l'articolo 2. Esprimo pertanto parere favorevole all'emendamento 5.19.

è abbastanza controverso: io personalmente milito a favore delle ragioni esposte dal collega Izzo. Il tema della vicedirigenza, che non può essere assolutamente dribblato anche in questa occasione,

5.9 il punto 3), che ci sembra troppo prescrittivo e restrittivo rispetto alle incompatibilità, mentre invece gli altri due punti potrebbero essere sicuramente considerati

ho chiesto al presidente Chiti, che ci aveva riferito di una precisa determinazione del Consiglio di Presidenza riguardo alle schede, se non dovessero essere tolte anche le schede che danno presente il senatore, pur senza dar luogo a votazione. Il presidente Chiti mi ha risposto: assolutamente sì. La pregherei quindi di far togliere anche le schede che, essendo inserite, segnano la presenza del senatore anche se non danno luogo ad espressione di voto. Invitiamo i senatori Segretari ad individuare quali siano le schede in

Prego, senatore

non per campanilismo, in quanto figlio di vecchio chirurgo ospedaliero, primario e pioniere della chirurgia che ha allevato generazioni di chirurghi, ma perché

anche gli aiuti ospedalieri o dirigenti di struttura semplice, come oggi si dice con linguaggio amministrativamente più moderno. Inoltre, onorevoli onorevoli colleghi, non possiamo disconoscere che nell'applicazione delle norme oggi le ASL stanno compiendo in tutta Italia (in qualche zona peggio) ogni sorta di discriminazione attuando trattamenti preferenziali, manco a dirlo, a seconda dei legami

o ai responsabili di incarichi professionali specifici e, quanto alla decorrenza, avrei preferito che, anziché al compimento dell'anzianità contributiva, si fosse fatto riferimento all'adozione del provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro per compimento dell'anzianità massima contributiva;

vorrei associarmi a quanto appena dichiarato dal senatore Benedetti Valentini con l'auspicio che questa norma possa essere estesa anche agli aiuti universitari e non solo ai primari.

ordine del giorno è infatti finalizzato al ridimensionamento delle *lobby* dei baroni universitari e della vera casta, quella dei magistrati, uniformandoli alle altre categorie del pubblico impiego. Mi rivolgo direttamente a lei, signor Ministro, considerando che ci accingiamo ad approvare un disegno di legge delega, affinché ella possa recepire il contenuto del citato ordine del giorno già nei decreti attuativi di questa legge, ponendo fine una volta per tutte ai privilegi delle *lobby*, delle caste quelle vere - dei magistrati e dei baroni universitari.

Non c'è dubbio che la materia della permanenza in servizio e delle deroghe ai limiti d'età va ripensata e riformulata alla luce di quanto accadrà sul piano pensionistico,

Repubblica, in seguito all'approvazione dell'emendamento 5.305 al disegno di legge n. 847, il Senato impegna il Governo a rivedere l'età pensionabile delle categorie di cui al comma 11 dell'articolo 72 della legge 6 agosto 2008, n. 133, uninformandone l'età pensionabile alle altre categorie del pubblico impiego».

Alla faccia dei giovani, di quanto si pensa di poter fare in termini di rinnovamento del Paese oltre che di assicurare un'età giusta per la pensione soprattutto per talune categorie.

a favore di questo ordine del giorno. Le critiche che sono arrivate finora dai senatori che mi hanno preceduto nel dibattito sono del tutto irricevibili, perché ormai da molti anni si assiste ad un Far West nelle Regioni sulle modalità di rapporto di lavoro in ordine al tempo e all'età. È del tutto pretestuoso cercare di dire che con questo si creerà una illegittimità, quando l'illegittimità è palese allo stato di fatto. ADAMO accelera la soluzione di un problema che voi non siete riusciti a risolvere per due anni. Quindi, noi siamo convintamente

Dichiaro aperta la votazione.

apprezzato un'iniziale disponibilità del relatore - come spesso è capitato - che ha accolto anche un nostro emendamento, poi però, come già hanno rilevato i colleghi, per il resto dell'articolo questa disponibilità non c'è più stata. Sono stati respinti degli emendamenti, da noi illustrati, che vanno esattamente nello stesso senso del primo, cioè che responsabilizzano in modo più preciso l'azione della dirigenza, dando dei poteri molto importanti per l'efficienza della pubblica amministrazione. Tre o quattro dei nostri emendamenti qualificanti sono stati inspiegabilmente così come quello sull'incompatibilità, che ci sembra in linea con i principi di moralità e di distinzione di cui stiamo tanto parlando.

Presidente, intervengo non per fare polemica, ma solamente per chiarire e poter migliorare il percorso dei nostri lavori futuri. Quando un ordine del giorno è accolto dal Governo, solitamente, per prassi, questo non viene messo ai voti. Vorremmo sapere se questa prassi da parte della Presidenza è confermata o meno. Detto questo, nessuna polemica su quello che è avvenuto.

la disciplina oggi vigente prevede che, quando un ufficio o struttura sia in situazione di grave sofferenza dal punto di vista dell'efficienza o produttività, sia dovere del dirigente provvedere alla rimozione di questa situazione fondamentalmente con la collocazione in *stand-by*, in mobilità dei dipendenti in eccedenza. di un provvedimento molto severo, molto rigoroso, che di fatto non viene mai adottato. Per questo motivo riteniamo che, senza

paralizzando gli aumenti retributivi in quella determinata situazione, anche al fine di consentire che si crei un incentivo per l'accettazione della mobilità verso strutture diverse. Questa è la soluzione che può aiutare a risolvere il problema. L'emendamento 6.4 mira sostanzialmente a questo,

Signora Presidente, signor Ministro, signori senatori, l'emendamento 6.0.12 attiene alla problematica della specificità delle forze militari e delle forze di polizia. Già sono state sottolineate, anche nella seduta odierna, la peculiarità e la particolarità dei compiti che il personale appartenente a tali forze è chiamato ad assolvere. È stato già evidenziato anche l'alto livello di efficienza espresso dal comparto della pubblica amministrazione che è composto proprio da quel personale, così come sono già stati posti in rilievo l'elevato consenso e la grande fiducia che l'opinione pubblica manifesta nei confronti dell'operato degli uomini e delle donne in uniforme. In aggiunta a ciò, non possiamo dimenticare come lo *status* del personale militare e di polizia sia legato all'assunzione e al rigoroso rispetto di doveri che gli altri dipendenti pubblici non hanno. non possiamo dimenticare come la lotta alla criminalità e la salvaguardia della sicurezza e delle istituzioni, a cui quelle forze sono preposte, comporti sempre un alto livello di rischio per gli appartenenti ad esse. Spesso, purtroppo, in Italia e all'estero quel personale ha pagato con gravi infermità permanenti o addirittura con la vita la sua dedizione al servizio e al bene del Paese. So che queste valutazioni e questi sentimenti sono condivisi dalla maggioranza dei senatori, che in più circostanze hanno esaltato il senso del dovere e i sacrifici delle Forze armate e di polizia. Ed è proprio su questa base che rinnovo all'Assemblea un invito pressante: diamo un segnale concreto di attenzione al personale militare e alle forze di polizia, attraverso la corresponsione di una indennità specifica, anche se di contenuta entità. Diamo questo segnale, ricordando che è quello stesso personale a cui le istituzioni e la gente si rivolgono ogni giorno e in particolare nei momenti più difficili della vita del Paese, certi di ricevere sempre

Non si comprende dunque perché una norma, già approvata dalla Camera dei deputati e che i relatori Saltamartini e Castro stanno portando avanti anche al Senato, dovrebbe essere inserita in questo provvedimento, che invece è in prima lettura e poi deve essere

Grazie non intendo ritirare questo emendamento. Ringrazio il senatore Vizzini per le sue precisazioni, che a me erano già note. Vorrei soltanto precisare a quest'Aula che i fondi attualmente previsti per per l'indennità per la specificità consentono di retribuire tutto il personale delle Forze armate e di polizia con l'imbarazzante cifra di tre euro al mese. Questo era l'intendimento dell'emendamento 6.0.12: cercare di evitare che quel personale (che naturalmente guarda al Parlamento) si vedesse ricompensato, per quello che fa, con tre euro al mese. Infine,

pertanto che esso debba essere rimodulato. Ecco perché prevedevamo la soppressione non già per negare il lavoro prodotto e dalla Commissione e dal relatore e dal Comitato ristretto, ma perché riteniamo che in questa proposizione sia dato spazio più alla contrattazione sindacale (e quindi al favoritismo) che non al riconoscimento del merito di ciascun dipendente.

firma. Vorrei invitare ad esaminare questo aspetto ed eventualmente a modificare l'articolo 7 così com'è stato proposto dalla Commissione.

Lo ha sostenuto, per almeno quattro anni, qualcuno che è ben più in alto di me nella gerarchia di partito e, se permettete, in questo momento anche nella gerarchia istituzionale parlamentare.

cancellandola dal nostro ordinamento. Con buoni intenti perveniamo ad un risultato perverso, rimettendo la questione ad una serie di contrattazioni di primo e di secondo livello per cui sarà vero tutto e il contrario di tutto. L'intento è quello di non applicare la legge

che i nostri emendamenti, che laconicamente propongono di sopprimere l'articolo 7, cercano una soluzione costruttiva di assoluta mediazione, di equilibrio. Ritengo che il Governo potrebbe accedere a questa nostra impostazione e che l'intera Aula potrebbe orientarsi verso un voto che verrebbe accolto come un segnale di ma certamente molto importante verso soluzioni cercate per tanti anni e che potrebbero, senza essere qui pregiudicate, aprirsi di qui ai mesi successivi dando al Governo il tempo, il modo e il quadro razionale per poter affrontare il problema. Questo è l'auspicio costruttivo che io e gli altri colleghi firmatari rendiamo all'Aula e ai colleghi del Governo.

utili all'Agenzia di valutazione, intervenire su fondi già stabiliti e sottrarli ad una destinazione già stabilita per legge.

della vicedirigenza. Mi sembra una proposta che possa contribuire a trovare una soluzione di sintesi per questa materia così fortemente attesa.

vorrei dire che questa è la prova del fatto che, se il suo testo originario fosse rimasto tale, lo spettacolo di un Parlamento che si occupa delle singole questioni corporative e di un pezzo del mondo del lavoro del pubblico impiego sarebbe diventato assolutamente devastante. Aver confermato invece la sovranità e le modalità della contrattazione, nonché la sovranità delle parti nella contrattazione credo che sia stata una operazione politica di grande rilievo che non fa tornare indietro le lancette a vent'anni fa, allorché la politica ne fece di tutti i colori nella gestione del personale della pubblica amministrazione, ma finalmente guarda avanti e conferma che la sovranità della contrattazione è quella che consente davvero di fare quel salto di innovazione che mi pare stia emergendo dal testo che stiamo discutendo.

Qui si sta trattando una norma di interpretazione autentica che rimette in discussione l'introduzione, da oltre sei anni, dell'area della vicedirigenza e lo si fa pagando un prezzo alle organizzazioni sindacali per non far uscire dal comparto e dalla contrattazione collettiva la parte più importante della pubblica amministrazione, che è sottoposta ad un criterio di disciplina e di valutazione pari a quello di altro personale pubblico di comparto, ma con qualifiche e professionalità inferiori. In realtà, segnalo una duplice incoerenza: da un lato - e facciamo bene -introduciamo il principio in forza del quale l'organizzazione della pubblica amministrazione e degli uffici ritorna in capo allo Stato attraverso la legge e, quindi, decontrattualizziamo questa parte del settore del pubblico impiego, cosa importante di cui va dato atto al ministro Brunetta. D'altro canto, affidiamo invece alla contrattazione la disciplina integrale, ivi compresa la riorganizzazione, di questa fascia di personale rappresentata dai quadri della pubblica amministrazione, che dovrebbero essere incentivati, perché non sono soggetti a *spoil* *system* e dovrebbero garantire il principio di imparzialità

questo articolo 7 sia politicamente vergognoso. Voteremo pertanto a favore della soppressione di questa norma, perché crediamo che sia una vergogna ed una mortificazione del personale statale e dell'amministrazione che lavora e che vuole essere valutata per ciò che fa, non per quello che dicono le organizzazioni sindacali.

mi rivolgo in modo specifico ai colleghi della maggioranza parlamentare, perché l'intervento fatto dall'esimio collega dai banchi dell'opposizione di sinistra è sintomatico.

tutto il provvedimento che il ministro Brunetta, il Governo e la maggioranza portano avanti è strutturato sulla logica di ridare certezza del diritto ed oggettività alle strutture, alle impalcature ed all'organizzazione dei quadri, per sottrarla all'arbitrio, alla partigianeria, alle superfetazioni sindacali e quant'altro. In questo caso, invece di ottemperare ed attuare una legge dello Stato, che prevede un certo livello per i quadri e che viene in un certo modo a rendere omogenea la pubblica amministrazione con i comparti privati, stabilendo per i quadri una disciplina parallela e omogenea, ebbene noi invece facciamo un salto all'indietro, non so in quale Repubblica, per stabilire che debba essere *ad* *libitum* della contrattazione sindacale il poter o non poter riconoscere certi diritti, non solo, ma il valutare certe funzionalità della struttura pubblica amministrativa. Scusatemi, questo non rientra nella logica informatrice del provvedimento portata avanti dal Governo, non è nello spirito del voto convergente che si è manifestato su molte norme anche nell'*iter* del provvedimento stesso

che lascia perlomeno la situazione legislativa vigente e non peggiora e non compromette la situazione, sia accolta. Sintomatico sul piano politico dell'attualità politica l'intervento del collega di opposizione; mi auguro che sia valso anzi a schiarire le idee a chi poteva eventualmente, con tutto il rispetto, non averle ben orientate. Insisto pertanto per la votazione di tale emendamento e voterò favorevolmente anche all'emendamento del collega Izzo.

Se fosse possibile, in via preliminare, invitare il ministro Brunetta al ritiro di un articolo del genere, lo farei volentieri. È noto a tutti che la Corte dei conti necessita sicuramente di una riforma, che deve però essere seria, approfondita e completa. Invece, quest'articolo 9 contiene al proprio interno delle norme in contraddizione tra di loro, norme insufficienti e sicuramente non organiche, tanto è vero che lo stesso relatore e mi pare addirittura un collega senatore della maggioranza propongono emendamenti che cercano di precisare un po' la situazione. Una riforma così incisiva delle competenze, della struttura e della stessa composizione dell'organo di vertice della magistratura contabile non si può realizzare con un mero emendamento ed un collegato alla finanziaria. Ciò per diversi motivi, non ultimo perché una così importante riforma delle attribuzioni e della struttura della Corte dei conti avrebbe richiesto, necessariamente, la previa consultazione dell'avvocatura, del mondo accademico ma, soprattutto, della magistratura contabile. Questa, invece, attraverso i suoi organismi, ha criticato in maniera abbastanza pesante la riforma in esame. Questa iniziativa normativa rischia d'intervenire pesantemente sulle funzioni e sull'ordinamento della Corte, in contrasto con le esigenze, con le garanzie poste dalla Costituzione a tutela del corretto utilizzo e della proficua gestione delle risorse finanziarie pubbliche, nonché con i principi posti a presidio delle magistrature. In particolare, è modificata la coerenza del sistema costituzionale di controllo esterno della Corte dei conti, controllo che verrebbe ad essere asservito e subordinato ai Governi centrali e locali; ciò, lo sottolineo, a detrimento del corretto rapporto con il Parlamento e con queste assemblee elettive. Il testo introduce, inoltre, principi e criteri gerarchici e accentratori, specie attraverso l'attribuzione al vertice dell'istituto di una funzione di indirizzo politico e istituzionale che è propria delle strutture burocratiche, ma che viene così estesa anche al governo delle funzioni magistratuali, in maniera che pare non compatibile con i richiamati principi costituzionali. Inoltre, appare lesivo delle attribuzioni dell'organo di vertice della magistratura contabile, il Consiglio di Presidenza, il pressoché totale annullamento, a vantaggio del solo Presidente, delle sue funzioni che ora si riducono a mansioni di mera amministrazione del personale di magistratura, ed è sostanzialmente per questo, ritenendo che sarebbe indispensabile una riforma organica della Corte dei conti, che viene proposto l'emendamento soppressivo 9.300.

completamente diverso rispetto a quella che è la Corte dei conti attuale, attribuendo ad essa ruoli e compiti inusitati e completamente diversi. Si alterano le funzioni della Corte dei conti e si prevedono nuovi e incisivi poteri di controllo sulle gestioni pubbliche e statali. In pratica, la Corte dei conti, in questa maniera, diventa un organo servente del Governo e io penso che una qualche autorità costituzionale si troverà, ad un certo punto, a misurare questo articolo e sarà costretta ad espungerlo, a renderlo inoffensivo.

su questo emendamento. Condividiamo perfettamente le ragioni che il collega Casson ha posto a base del suo emendamento, ma vogliamo sottolineare con la nostra astensione l'assoluta necessità che si provveda quanto prima ad una seria riforma della Corte dei conti. Alcuni dei principi che sono contenuti nell'articolo 9, in realtà, sono condivisibili e altri no, ma già nella scorsa legislatura avevamo presentato emendamenti in questo senso. Quindi, pur comprendendo perfettamente le ragioni del collega Casson, il collega Marini ed io ci asterremo perché vogliamo segnalare che

l'articolo 9 debba essere soppresso. State facendo un grande errore: non si può riscrivere l'ordinamento e l'esercizio delle funzioni autonome della Corte dei conti e del Consiglio di Presidenza mediante

9 si parla di effettuare controlli sulle gestioni pubbliche e statali in corso di svolgimento, il che non si comprende che cosa tecnicamente significhi. È un controllo di gestione? Allora, introduciamo una norma che disciplini il controllo di gestione. È un controllo concomitante? Allora, rivisitiamo il sistema dei controlli concomitanti della Corte dei conti. Che cosa è? Che tipo di controllo è? Come viene esercitato? Su quali atti? Sul procedimento? Sull'impegno di spesa?

che se vengono individuate gravi irregolarità gestionali, ovvero gravi deviazioni da obiettivi, procedure o tempi di attuazione stabiliti dalle norme, la Corte ne individua le cause in contraddittorio con l'amministrazione. Ma se vengono accertate gravi irregolarità gestionali siamo in presenza di un illecito erariale e, quindi, dell'accertamento del danno che produce, come unico effetto, l'esercizio dell'azione di responsabilità amministrativa e contabile

il problema è quello dello snaturamento di una funzione costituzionale principale, che viene meno. Noi stiamo discutendo nell'ambito della riforma della giustizia se creare uno o più CSM o se accorpare in un unico CSM tutte le funzioni e tutte le magistrature, e voi, con un colpo di emendamento, venite qui a modificare il consiglio superiore che si occupa della magistratura contabile? Siamo veramente impazziti? È veramente una follia! Tornate indietro su questo articolo!

Signora Presidente, da lunedì le cronache locali e regionali del Paese ci parlano di un vero e proprio bollettino di guerra. Le Regioni Lombardia, Veneto, Liguria, Toscana e Trentino-Alto Adige, solo per citare quelle che sono intervenute in maniera più eloquente, hanno manifestato in termini sempre più vibranti la loro denuncia di disservizi,

Riteniamo pertanto assolutamente urgente che il Ministro competente venga a riferire in Parlamento sullo stato di disagio ampiamente rappresentato. rappresentato. Troviamo inaccettabile che i costi di attivazione di una infrastruttura fondamentale per l'ammodernamento del Paese, e che ci vede convinti sostenitori, siano scaricati a danno degli utenti più deboli, soprattutto pendolari, lavoratori e studenti. Allo stesso modo, troviamo insopportabile lo scarico di responsabilità, ancora oggi rappresentato nelle cronache e sulle agenzie di stampa, fra Regioni e Ferrovie dello Stato sulla mancata copertura dei servizi regionali e dei treni a lunga percorrenza. Signora Presidente, ci rivolgiamo pertanto a lei e per suo tramite al presidente Schifani, affinché con la sua autorevolezza, anche in ragione dell'importante incontro che avverrà domani tra il Ministro e le Regioni per il riparto dei 480 milioni assegnati al trasporto pubblico locale e ai servizi regionali ferroviari, chieda al Governo di venire a riferire subito in Parlamento per mettere un punto fermo sullo stato dell'arte circa la situazione che così diffusamente si è determinata nel Paese - lo voglio ricordare ancora una volta - riguarda le condizioni di vita e di lavoro di milioni di nostri concittadini. Confido, ovviamente, nell'interessamento attento e sensibile della Presidenza e, in particolar modo, del presidente Schifani.

Grazie